L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, come preannunciato ai Gruppi per le vie brevi, comunico che, sulla base del calendario corrente, la relazione sull'amministrazione della giustizia sarà svolta dal ministro Alfano nella seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 16.

13,59)*. *Allegato A* DISEGNO DI LEGGE Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

avendolo utilizzato in gran parte per discutere sulla rilevantissima questione del rinvio in Commissione degli emendamenti del relatore e dei relativi subemendamenti.

che la scansione temporale della conclusione di questo provvedimento consente certamente l'utilizzo di un ulteriore spazio temporale e che stiamo per affrontare il grosso degli emendamenti e dei subemendamenti in alcun modo - come ci è noto - esaminati dalla Commissione di merito; abbiamo, assoluta necessità di discutere ed interloquire su di essi e, ovviamente, anche sugli altri. Il secondo tema riguarda l'emendamento accantonato 1.0.1002. Ricordiamo tutti che questo emendamento fu accantonato la settimana scorsa soprattutto in rapporto alla lettura dello stesso e alla norma transitoria di cui al successivo emendamento

relativamente al regime transitorio. Volevo sollecitare e porre formalmente, eventualmente con riserva di esame, la proponibilità da parte nostra dello stralcio dell'emendamento del relatore e, quindi, dei relativi subemendamenti. Non sfugge

su una materia del tutto nuova. Questo emendamento - la cui forza è evidente, provenendo dal relatore - non è stato in alcun modo esaminato, come ci è noto, dalla Commissione di merito e, quindi, crediamo che possa essere adottata una decisione

ove non si accedesse all'interpretazione estensiva che ho proposto, si determinerebbe una chiara violazione di una delle prerogative riservate ai singoli senatori e ai Gruppi. Ecco perché le sollecito l'esame di tale questione e una decisione in tempi ragionevoli e ristretti, in modo tale da poter esercitare questa prerogativa.

Signor Presidente, formulo la mia richiesta e intervengo adesso, prima ancora che sia assunta la decisione sull'istanza formulata dal senatore Legnini, per evidenti ragioni di economia di gestione dell'attività parlamentare. Sarò molto breve. Tutti i poteri, vieppiù quello della rappresentanza popolare e della produzione dei provvedimenti legislativi, devono essere caratterizzati dal massimo della trasparenza. Circolano non so quanto fondate, e questa è la ragione della mia richiesta - le voci più varie sulla possibile applicabilità della norma, di cui vi ha ora parlato

alla discussione di questo emendamento il Governo ci dica se ha valutato la sussistenza di tali condizioni e se effettivamente è vero - come si adombra da più parti - che vi sarebbero appartenenti al Governo o ai Governi passati e alla maggioranza presente che verrebbero a beneficiare anche soltanto della norma nella sua riformulazione. In sostanza,

di parlare con alcuni magistrati della Corte dei conti per verificare la compatibilità dei termini fissati da questo emendamento sul processo breve, chiedendo quali sono i tempi di celebrazione oggi presso la Corte dei conti: ebbene, mi hanno detto che i termini erano corretti.

ma non possiamo aprire un dibattito in fase preliminare. Lei si è espresso, le è stato risposto; interverrà quando si arriverà a questo emendamento.

Presidente, se la sua comunicazione deve intendersi come un rigetto dell'istanza che ho avanzato, comunico che non accettiamo la decisione presa e ci riserviamo di riproporla al momento della

Colleghi, da parte dei senatori Legnini ed altri sono state presentate 78 richieste di voto segreto su emendamenti e subemendamenti agli articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame. La Presidenza ha valutato queste richieste alla luce dei criteri che informano in via generale l'ammissione di articoli ed emendamenti al voto segreto, criteri già comunicati all'Assemblea nella seduta del 24 marzo 2009, che si ritiene opportuno ribadire anche in questa sede. Ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento «l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano» e comunque in modo palese. La modifica regolamentare del 1988 fu dettata dall'intento di «circoscrivere a casi rigorosamente determinati l'area del voto segreto», che pertanto «non può essere ammesso per tutte le deliberazioni che implichino un generico riferimento ai diritti di libertà» richiamati dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, «ma solo per quelle che abbiano per effetto la limitazione o la compressione dei diritti stessi». Le richieste avanzate dai senatori Legnini ed altri si possono sinteticamente ricondurre a sei tipologie principali: modifica ai termini - e ai casi di sospensione dei termini - di ragionevole durata delle fasi di giudizio, il superamento dei quali comporta l'estinzione del processo secondo l'impianto del disegno di legge in esame; modifiche alla disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni ai fini della certezza dei tempi e dell'efficienza del sistema giudiziario. *(Brusìo)*. Colleghi, o c'è silenzio in Aula o sospendo la seduta.

modifiche alla disciplina sanzionatoria per determinate fattispecie di reato, tendenti all'innalzamento del massimo della pena oltre il limite dei dieci anni al fine di determinare l'esclusione dalla proposta disciplina sull'estinzione del processo. I proponenti fondano prevalentemente le proprie richieste sui princìpi costituzionali di «libertà personale, tutela giurisdizionale dei diritti,

alla finalità di adeguare il processo penale, nelle sue diverse fasi, ai principi del "giusto processo" richiamati dall'articolo 111 della Costituzione, con particolare riguardo alla "ragionevole durata" di cui al secondo comma. I diversi ed articolati principi ricavabili da tale norma costituzionale - che non rientra tra quelle indicate dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, quale presupposto per eventuali richieste di votazioni a scrutinio segreto appaiono nel loro insieme prevalenti rispetto al richiamo effettuato dai proponenti ai principi costituzionali individuabili, ancorché non espressamente indicati, negli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione. Pertanto, la Presidenza non ritiene di poter ammettere allo scrutinio segreto gli emendamenti e subemendamenti rientranti in tali categorie. Diverso è invece il caso degli emendamenti tendenti ad apportare modifiche al codice penale in materia di prescrizione e disciplina sanzionatoria di determinati reati che, per la loro natura sostanziale e non meramente processuale, la Presidenza considera riconducibili ai principi costituzionali relativi alla libertà personale e al principio di legalità di cui agli articoli 13 e 25 della Costituzione, nonché alla tutela della famiglia ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione. Pertanto potranno effettuarsi votazioni a scrutinio segreto sui seguenti emendamenti: - in materia di prescrizione: 2.1000/31 (pag. 187); 2.1000/33

in materia di disciplina sanzionatoria di reati: 2.0.7 (pag. 297); 2.0.10 (pag. 298); 2.0.45 (pag. 298). È in distribuzione ai Gruppi l'elenco degli emendamenti ammessi allo scrutinio segreto.

Presidente, noi proponiamo la soppressione dell'articolo 2. Le ragioni di questa nostra richiesta sono state esplicitate in più circostanze anche se - ahimè - l'Aula, soprattutto nella sua maggioranza, sembra, più che sorda, distratta e disinteressata agli argomenti che abbiamo esplicitato in maniera serena, chiara e costruttiva. L'articolo 2, anche nella versione

una previsione di durata, un termine entro il quale lo Stato debba o possa esercitare il suo potere-dovere di reagire alle aggressioni criminali o, comunque, di dover decidere su istanze dei cittadini. La prescrizione del processo è innaturale, è dannosa, è, così come introdotta da questo disegno di legge, che noi temiamo possa tramutarsi in pochi giorni in legge vera e propria, qualcosa che non solo stride con l'intero sistema italiano, italiano, ma che cozza in maniera quasi offensiva con le dichiarazioni o con la presentazione di questo disegno di legge. La prescrizione del processo non ha ragion d'essere perché l'obiettivo principale di uno Stato di diritto è quello di espletare i processi, che sono uno strumento ineliminabile per accertare la verità. Questo è un valore riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione. Intervenire a fronte di un di un eccesso di tempo, di un tempo irragionevole, che oggi registriamo in quasi tutti i processi, dicendo che questi si estinguono decorso un certo periodo, senza fare nulla questo è il punto cruciale: ripeto, senza fare nulla - perché i processi possano obiettivamente essere celebrati in tempi ragionevoli, significa non voler risolvere i problemi; significa mentire in maniera grave, là dove scrivete:

Il collega Maritati ha illustrato molto bene le ragioni per cui chiediamo la soppressione dell'articolo 2, destinato a creare dei disastri all'interno del sistema processuale penale.

Mi limito ad indicare soltanto i temi sui quali interveniamo, partendo proprio dall'emendamento 2.1000/28: si fa riferimento ad interventi e a disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del procedimento; si cerca di intervenire sul processo telematico, sugli archivi informatizzati, sul cosiddetto processo *in absentia*, sul rito degli irreperibili

ciò per dare il senso politico, concreto e positivo della nostra opposizione. Prendiamo però atto, ancora una volta che, come in Commissione, probabilmente anche in quest'Aula otterremo una risposta negativa.

rispetto alla decadenza dei processi, il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Al di là delle considerazioni di ordine generale che si possono avanzare sul tema della priorità e della gerarchia dei reati, per cui nel primo testo non si considerava il mio emendamento era stato sollecitato dal Consiglio comunale di Milano nella sua interezza.

a tutta l'Assemblea questo problema, che ha ovviamente risvolti di ordine generale, ma che per Milano presenta una sua specificità, che tradotta in soldi vuol dire 100 milioni di euro che rischiano di essere sottratti

Presidente, il tema è stato ampiamente trattato nel corso del dibattito; anche durante la riflessione ulteriore che il Presidente del Senato concesse in Commissione proprio per discutere di questi argomenti, prima che venisse meno l'ipotesi di dialogo auspicata, c'era stata una relazione da parte dal relatore su questi temi. L'articolo 2 è finalizzato a razionalizzare ulteriormente il testo che faceva parte del documento legislativo originario. Si sono escluse quelle ipotesi per le quali la ragionevole durata del processo, prevista dall'articolo 111 della Costituzione, non dovesse essere applicata a soggetti a soggetti che avessero precedenti penali, quasi che i tempi del processo debbano essere diversi a seconda che un soggetto abbia avuto o meno pregresse esperienze. L'obbligo dello Stato di condurre il procedimento entro i tempi previsti dalla norma costituzionale deve valere per tutti e verso questo criterio verso questo criterio ci si è orientati eliminando quelle ipotesi che erano contenute nel disegno di legge ordinario. Analogamente è apparsa è apparsa incoerente, o forse irragionevole rispetto al dettato costituzionale la possibilità che la ragionevole durata afferisse soltanto ad una determinata tipologia di reati, di reati, quelli la cui pena era contenuta entro i dieci anni di reclusione, e venissero esclusi una serie di altri reati che suscitavano particolare allarme sociale.

salvo alcune peculiarità che determinerebbero una ricerca del particolare che andrebbe poi a confliggere con l'esigenza costituzionale - meno grave di un

Così come per una fascia dei reati che suscitano particolare inquietudine e allarme sociale - cito, per brevità, soltanto quelli relativi alla mafia e al terrorismo - si impongono tempi di valutazione assolutamente diversi, più congrui ed adeguati alle difficoltà ed alle complessità che le indagini comportano. Quindi, questi sono i principi ai quali il relatore si è ispirato. Naturalmente è prevista è prevista una serie di ipotesi ulteriori che afferiscono alla sospensione del termine nel momento in cui si svolgono talune attività. principio contenuto nell'emendamento del relatore appare assolutamente coerente con il dettato costituzionale, un'esecuzione corretta del precetto di cui all'articolo 111

consentiva ai capi degli uffici di sospendere i processi che presumibilmente avrebbero beneficiato dell'indulto per un termine non superiore a 18 mesi; siccome vi è una norma transitoria in questo provvedimento, ci è sembrato quanto mai singolare immaginare che sia l'estinzione del reato - decorsi i termini previsti dalla nuova formulazione dell'articolo 2 - sia l'ipotesi della norma transitoria potessero beneficiare anche dell'ulteriore sospensione prevista dal decreto‑legge n. 92 del 2008. Per questa ragione quel termine non viene computato

portato. L'introduzione del processo breve, volto a disincentivare l'ingiustificata inerzia dall'autorità giudiziaria, è ovviamente un obiettivo di civiltà sul quale

Occorre però che questo risultato venga perseguito innanzitutto attraverso l'uso di criteri razionali ed equi, tassativi ma anche elasticamente modellabili sul caso concreto; necessario riportare l'elefantiaco sistema penale alle sue dimensioni minime, o almeno - nel breve periodo - predisporre meccanismi trasparenti, controllabili e democratici di selezione delle iniziative accusatorie. L'attuale disegno di legge, invece, fissa brutalmente, dall'oggi al domani, sull'onda dell'ennesima emergenza strumentale, scansioni temporali totalmente irrealistiche se commisurate al numero di procedimenti pendenti, il che non può che aumentare il tasso di ingiustizia, di arbitrarietà e di antidemocraticità del processo penale, abbandonando definitivamente le vere scelte sui tempi agli incontrollabili particolarismi dei singoli uffici giudiziari o, peggio ancora,

Il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame risulta, al tempo stesso, irragionevole ed inefficace in quanto agisce esclusivamente sulla determinazione della durata massima delle singole fasi processuali, senza sanzionare con analogo meccanismo la durata eccessiva della fase procedimentale delle indagini preliminari. Spesso infatti si verificano inammissibili ritardi nell'esercizio dell'azione penale, con il conseguente determinarsi di lunghissimi tempi morti fra effettiva conclusione delle indagini ed esercizio dell'azione penale. Gli emendamenti in questione pertanto tendono a sanzionare anche la durata eccessiva delle indagini preliminari, prevedendo nel contempo l'introduzione di una norma che preveda la responsabilità disciplinare del pubblico ministero titolare delle indagini nel caso si verifichi una eventualità del genere. Dichiaro il voto favorevole anche a nome della senatrice Poretti.

che per la fase dell'appello che, salvo ipotesi di parziale rinnovazione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, si risolve nella maggior parte dei casi in una sola udienza di discussione. Pertanto con l'emendamento 2.1000/16 la Pertanto con l'emendamento 2.1000/16 la durata del giudizio di secondo grado si ridurrebbe da 24 a 18 mesi. Inoltre appare più ragionevole far decorrere il termine riservato al giudizio d'appello non dalla redazione della sentenza emessa nel grado precedente, ma dal deposito dell'atto di impugnazione, in modo cioè che i periodi fisiologici necessari alla redazione della sentenza, che possono essere anche di 90 giorni, e quelli riservati all'esercizio del diritto di impugnazione, che possono arrivare fino a 45 giorni, non sempre decorrenti dalla scadenza del termine anzidetto, non vengano computati ai fini della dichiarazione di estinzione del processo.

perché valgono per la fase successiva, relativa al giudizio di legittimità, per il quale neppure vale la possibile eventualità della rinnovazione istruttoria. Anche in questo caso, dunque, la previsione di una durata di fase di due anni appare del tutto irragionevole in sé e del tutto sproporzionata rispetto a quella prevista per la fase dibattimentale. Di qui, secondo noi, la necessità di ridurre il termine da 24 a 18 mesi prevista anche con l'emendamento che - ahimè - farà la stessa fine, avendo ancora una volta dovuto ascoltare i pareri contrari anche a tutte quelle minime misure di miglioramento di un testo che tutto vorrà fare tranne che aiutare l'amministrazione della giustizia. Inoltre, come per l'appello, secondo noi appare più ragionevole far decorrere il termine riservato al giudizio di cassazione non dalla redazione della sentenza emessa nel grado precedente, bensì dal deposito del ricorso; ciò, in modo che i periodi fisiologici necessari alla redazione della sentenza stessa e quelli riservati all'esercizio del diritto di impugnazione non vengano computati ai fini della dichiarazione di estinzione del processo.

relativo ai procedimenti di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione. In questi casi, infatti, il disegno di legge prevede il termine di un solo anno, per cui il giudice deve dichiarare estinto il processo se, entro tale termine, non è stata pronunciata sentenza irrevocabile. Tenendo conto che le sentenze di rinvio sono comunque ricorribili per Cassazione, non si comprende come possa concentrarsi, in tale esiguo termine, il doppio grado di giudizio di rinvio e ricorso, o se debba scattare un ulteriore termine di fase tutto da identificare. Con questo emendamento si intende prevedere un termine di fase più lungo (due anni) per ovviare ai predetti inconvenienti.

dichiarazione di voto. Stiamo discutendo della giustizia penale nel nostro Paese e del fatto che il sistema viene completamente sconvolto. Noi non abbiamo nessuna intenzione di contribuire ad un provvedimento che distrugga la giustizia. Vorremmo che i cittadini avessero ben presente

colleghi, il voto segreto, quando richiesto e ammesso, come in questo caso, consente l'espressione a voto segreto del parere dei senatori; quindi non c'è una vittoria o una sconfitta: è del tutto

Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e del relatore su questo emendamento, che è sostanzialmente di forma, ma che può avere delle ricadute a livello interpretativo. L'emendamento 2.1000 del relatore,

e *c)*, ma viene pretermessa la lettera *d)*; quindi manca un ulteriore termine di un anno.

Io ho proposto di fare un riferimento specifico alle lettere, proprio per ovviare a qualsiasi difetto interpretativo. E poiché nell'ipotesi di reati particolarmente gravi (mafia e terrorismo) abbiamo aumentato il primo termine da quattro a cinque anni, il secondo da due a tre anni e il terzo da un anno e sei mesi a due anni, ho previsto che, per ogni grado di giudizio successivo alla sentenza di rinvio della Cassazione, anziché un anno si preveda un anno e sei mesi. Se il relatore e il Governo non ritengono di aumentare questo ulteriore termine da un anno ad un anno e sei mesi, per quanto mi riguarda sono d'accordo; però sono meno d'accordo sul fatto che vengano eliminate le specificazioni di cui ho parlato,

che in un Paese come il nostro si possa presentare da parte di una maggioranza di Governo un disegno di legge con un'intestazione menzognera, diretta a far credere al popolo che si intenda offrire uno strumento idoneo a ridurre i tempi notoriamente "irragionevoli" dei processi di ogni natura, mentre in realtà la legge, se tale diverrà, ha il solo scopo di impedire che uno o più processi pendenti a carico del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere comunque celebrato, un obbiettivo che consideriamo scellerato, non solo e non tanto perché il fine di rendere immune dal controllo giudiziario una persona costituisce una grave violazione del dettato costituzionale, ma soprattutto perché in questo caso si intende perseguire tale obiettivo attraverso una legge che avrà come conseguenza un'ulteriore destabilizzazione dell'intero sistema della giustizia nel nostro Paese. L'effetto della legge sarà in sostanza quello di impedire ad un numero indefinito ed indefinibile di processi di pervenire a conclusione, per via di un istituto assurdo che si introduce con la prescrizione del processo: un istituto inefficace e pericoloso, cui noi siamo decisamente contrari! Vorrei ricordare - ricordatelo anche voi - che uno dei compiti essenziali dello Stato di diritto è è quello di garantire la celebrazione dei processi, e non di decretare la loro estinzione a tempo, senza garantire la loro normale espletabilità! Invece, all'ultimo momento il relatore interviene

con un'eccezione che svela in modo definitivo lo scopo reale e scellerato del disegno di legge. Illustre relatore, l'allungamento dei termini di prescrizione e l'inclusione di tutti i reati e per tutti gli imputati in questo sistema perverso previsti dal suo emendamento, lungi dal limitare i danni, li aggrava perché coinvolge nel deleterio sistema della prescrizione dei processi tutte le materie processuali, tutti i reati, e nei confronti di tutti non riesco a vedere in cosa questa modifica potrebbe essere migliorativa rispetto al testo originario e a proposito di cosa. Si ostina il relatore a spiegare la bontà anche di tale correzione, ma non si vuol comprendere il grave errore di fondo. Prima è necessario creare le condizioni essenziali atte a consentire la celebrazione dei processi in tempi ragionevoli - certo, è questo un dovere impellente che incombe su noi legislatori -, poi si pretenda dagli operatori della giustizia il rispetto dei tempi,

Se comunque si dilata il termine di prescrizione entro i limiti che attualmente vengono consumati dalla gran parte dei tribunali, anche se non per tutti i processi, allora sorge spontaneo chiedersi (e ve lo a cosa serve questa legge, atteso che tutto deve restare come prima? La risposta la si trova con sorprendente chiarezza nella norma transitoria che chiude lo scellerato disegno di legge. infatti, fa un'eccezione alla dilatazione dei tempi di prescrizione - come modulati dall'emendamento del relatore - con riferimento ai processi penali di una certa fascia, che rientrino in un certo arco temporale, che poi evidentemente è quello in cui si trova collocato il processo a carico del Presidente del Consiglio dei ministri. Non vi sono parole che consentano di manifestare lo sdegno di tutti coloro che continuano comunque a credere in uno Stato di diritto! All'inizio dell'esame del disegno di legge abbiamo seriamente dichiarato la nostra disponibilità ad offrire proposte idonee a migliorare il testo mediante la previsione di interventi strutturali atti a garantire un'obiettiva contrazione dei tempi processuali. Abbiamo in sintesi proposto proposto la modifica urgente della geografia giudiziaria, che comporti la soppressione di un numero rilevante di sedi giudiziarie inutili e dannose, come riconosciuto e reclamato da tutti; l'introduzione dell'ufficio per il processo, atto a razionalizzare e velocizzare il lavoro dei magistrati; l'adozione del sistema integrato giudiziario informatizzato, già definito e pronto da realizzare sin dalla fine della scorsa legislatura; l'assunzione urgente di 2.800 cancellieri, senza i quali la gran parte degli uffici giudiziari continua a non poter funzionare, se non a ritmi inferiori ad ogni sia pur minima ragionevolezza. Tutte Tutte queste cose voi le sapete. Abbiamo chiesto, infine, l'adozione di alcune modifiche al codice penale che sono all'esame della Commissione e che in tempi brevi potremmo affrontare. A fronte di una generica disponibilità espressa dalla maggioranza, tutti i nostri emendamenti costruttivi sono stati bocciati anche dopo che la Commissione affari costituzionali - rammentatelo questo, perché è passato in sordina - aveva espresso un parere favorevole al testo di legge e agli emendamenti, condizionato ad alcune osservazioni, tra le quali la necessità di adottare tutti gli emendamenti che avessero come obbiettivo la predisposizione di interventi strutturali idonei a rendere possibile in concreto la contrazione dei tempi del processo (cioè quanto

Signor Presidente, ovviamente farò delle osservazioni di natura tecnica e mi rivolgo al relatore, presentatore dell'emendamento 2.1000, e al Governo. La scelta di fondo di questo emendamento è quella di aver collegato la gravità del reato alla durata del processo: ma questo è un criterio che è stato applicato, ed è in vigore, per quanto riguarda la prescrizione del reato; noi stiamo invece parlando di prescrizione dell'azione. E allora il medesimo criterio, gravità del reato ‑durata del processo, non tiene conto della, ma prescinde dalla complessità del processo.

Ha preso in considerazione, signor relatore, l'ipotesi in cui la Cassazione annulli con rinvio anche l'udienza preliminare, sicché in quell'anno dovrà svolgersi l'udienza preliminare e il dibattimento? Ha preso in considerazione tale Secondo punto. Lei prevede un termine di tre anni qualora venga esercitata l'azione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Qualora l'azione non venga esercitata in quei termini, comunque prevede che quei tre anni decorrano da due anni e tre mesi, cioè dal termine di durata delle indagini, ossia dal termine indicato dall'articolo 407: diciotto mesi, in caso di proroga, o due anni. Ha preso in considerazione l'ipotesi in cui, scaduto il termine delle indagini, l'indagato eserciti il diritto ai sensi dell'articolo 415-*bis*

Ha preso in considerazione l'ipotesi in cui, alla scadenza del termine delle indagini, il pubblico ministero chieda l'archiviazione,

di approfondire l'esame; presenti un testo tecnicamente accettabile e non contrassegnato da queste gravi irragionevolezze, quelle che le avremmo segnalato in Commissione giustizia se ci fosse stato consentito di lavorare in sede referente. Voteremo contro il suo emendamento o comunque le chiediamo una pausa di riflessione, un accantonamento per meglio modulare

Signor Presidente, non abbiamo difficoltà a riconoscere alcune questioni, sollevate nel corso del dibattito in Commissione, sono state, ancorché molto parzialmente, recepite in questo maxiemendamento del relatore, con riferimento ovviamente alla prescrizione del processo penale. Mi riferisco in modo particolare alla eliminazione di quella circostanza che rendeva obiettivamente incostituzionale il testo, in considerazione di una diversa applicazione della durata del processo a seconda della qualità soggettiva dell'imputato, cioè che fosse recidivo o no. Abbiamo affrontato tecnicamente il problema in Commissione e la questione della recidiva - che ha una sua complessità anche dal punto di vista processuale, oltre che da quello della sua preliminare gestione amministrativa - non avrebbe garantito la certezza dell'applicazione della norma ai soggetti con riferimento proprio all'accertamento della qualità Ciò detto, e preso atto anche della circostanza che si è tenuto conto, con riferimento al giudizio di primo grado, di di un allungamento dei tempi in considerazione della obiettiva durata di un processo penale in primo grado, dobbiamo dare atto al relatore anche per quanto riguarda la durata dei giudizi di rinvio. Ci permettiamo però di osservare, al di là delle considerazioni di carattere generale, che il testo che scaturisce da questo testo che scaturisce da questo dibattito, che nella sostanza è quello proposto dal collega Valentino, elimina alcuni profili di irragionevolezza e di incostituzionalità, ma rischia di introdurne altri. ad esempio, alla circostanza della estensione della prescrizione processuale anche alla fase delle indagini preliminari senza che quella fase

nella disciplina sulla prescrizione del processo penale ci sembra un rimedio peggiore del male, che non affronta il tema della durata delle indagini nella loro complessità, tema che la maggioranza aveva ritenuto di escludere dal dibattito parlamentare e dalle proposte emendative. Ora, introdurre un piccolo pezzetto di una disciplina nell'ambito della prescrizione del processo penale ci pare obiettivamente un fuor d'opera che rischia di complicare anche l'attività dei pubblici ministeri nel corso delle indagini preliminari. Il secondo aspetto che a noi sembra obiettivamente incongruente riguarda in modo particolare ciò che prima anche il collega Li Gotti ha sottolineato: il collegamento della durata del processo alla gravità del reato, senza tener conto della complessità del processo (e quindi del riferimento eventuale a più imputati e così via), rischia anche in costituire di fatto una disparità di trattamento nel processo applicando una regola generale a processi che, ancorché riguardino il medesimo reato, hanno una loro articolazione e una loro complessità totalmente diverse. L'unico elemento identico può essere il perseguimento di un determinato reato, ma ciò di per sé non rende uguali i processi nei quali si procede per il medesimo reato, perché vi possono essere processi che hanno più parti, e quindi hanno una loro complessità molto più ampia, e processi che viceversa sono di semplice e pronta definizione. L'altra questione che da alcuni punti di vista ci lascia perplessi è quella di aver inserito, nella discussione che riguarda la prescrizione processuale, alcuni processi che hanno un livello di allarme sociale estremamente elevato. Non v'è dubbio che l'ampliamento del tempo concesso può in qualche modo compensare l'attrazione in questa disciplina di processi che riguardano la mafia, il terrorismo, la riduzione in schiavitù o l'associazione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti,

che un'analisi dell'impatto di questa disciplina sui procedimenti in corso e sui futuri processi avrebbe consentito, e per la verità non ci è stato consentito perché discutiamo di questo emendamento in Aula e non abbiamo avuto la possibilità di farlo in Commissione), nonostante i limiti del dibattito e il contenimento oggettivo dello stesso in ragione di ciò che è stato proposto dal relatore e dalla maggioranza, ciò che obiettivamente rende indigesto il testo che ci accingiamo a votare è la sua applicazione ai procedimenti penali in corso.

che stiamo affrontando, o tentiamo di affrontare, una discussione sulla ragionevole durata del processo e non altro tipo di discussione che, secondo la nostra prospettiva e la nostra proposta politica, per quanto piccola e insignificante possa apparire, dovrebbe essere sviluppata in una sede diversa e propria, in linea con il dettato costituzionale. Faccio riferimento ovviamente al legittimo impedimento. Non è indifferente la circostanza che questa disciplina valga non solo per il futuro, ma anche per il presente: valga per il presente con una norma transitoria che, ancorché abbia ridotto l'impatto l'impatto della disciplina ai processi in corso, è comunque una norma incostituzionale, dal nostro punto di vista, che rischia di creare ancora più complicazioni estendendo l'indulto. Sarà simpatico vedere come i colleghi della Lega, che tanto hanno strillato contro l'indulto, voteranno questa norma transitoria che di fatto crea una coda dell'indulto tanto vituperato dalla Lega nella passata legislatura: sarà una cosa simpatica, sulla quale avremo modo di divertirci anche noi un pochino.

o saranno condotti fuori per le visite mediche, con aggravio di spese e oneri per lo Stato, per il personale e per loro stessi, oppure non saranno curati.

visto denunciato o fermato il loro contratto. Il tempo passato, dunque, non è molto, ma la contingenza è immediata e assoluta. Dobbiamo rispondere a più di 200 giovani ricercatori di alto livello

Se verrà una celere risposta del Governo, per pura contingenza risponderemo all'assemblea cittadina svoltasi venerdì scorso.

dell'influenza e gli sperperi e gli sprechi di un contratto sottoscritto dal nostro Ministro della salute, le cui clausole sono chiaramente vessatorie e sono sotto scrutinio della Corte dei conti. Un patto leonino che fa rimettere allo Stato, quindi a tutti i cittadini, qualcosa come 274 milioni milioni di euro a favore dell'industria farmaceutica Novartis. Mi chiedo come sia possibile che si possano sottoscrivere accordi, patti leonini, che penalizzano

prodotta da se stessa (sono loro che hanno prodotto l'allarme, che hanno condizionato l'Organizzazione mondiale della sanità; non so se verranno accertati anche reati di corruzione, staremo a vedere)

Riagganciandomi alle tematiche sollevate dal senatore Di Giovan Paolo relativamente all'immigrazione, desidero informare che in queste ore a Caserta è in corso un presidio non violento davanti alla prefettura. Come è noto, da Caserta provengono molti dei braccianti che a Rosarno sono stati al centro degli attacchi all'inizio dell'anno, braccianti che sono in Italia talvolta anche dall'inizio degli anni '90, molto spesso con permesso di soggiorno, valido o scaduto. Abbiamo avuto nelle settimane scorse, insieme al segretario Gaoussou Ouattara, un incontro con il ministro Brunetta per chiedergli che vengano rispettati i termini di legge: 21 giorni sono necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno, 21 giorni vengano utilizzati. Qualora vi fossero problemi amministrativi - chiaramente in Italia la burocrazia non si fa mancare nulla dal punto di vista dell'inefficienza - si adotti il silenzio-assenso, proprio per evitare di creare condizioni in cui, specie laddove lo Stato non è necessariamente presente, alla mancanza di una presenza di ordine pubblico si aggiunga la condizione di chi da legale si trova ad essere illegale, quindi alla mercé di organizzazioni criminali o informali per la raccolta stagionale di pomodori o arance.

Senatore Perduca, il suo intervento mi pare sia un richiamo all'applicazione della legge. Se poi ci sono ulteriori questioni, come quella relativa al silenzio assenso,

La permanenza del presidio dei Vigili del fuoco è necessaria perché ancora devono essere posti in essere interventi di messa in sicurezza di edifici, per la copertura degli stessi, per il recupero dei beni e delle masserizie. Si tratta di operazioni che ben difficilmente possono essere eseguite da altri soggetti che non siano i Vigili del fuoco. le notizie in possesso dell'amministrazione comunale di Marsciano risulta che il presidio straordinario è previsto solo fino al 24 gennaio. È quindi necessaria

In Sicilia non si vota per il rinnovo del Parlamento siciliano e non si vota in moltissimi Comuni: ecco perché registriamo il disinteresse del Governo nazionale rispetto a questa vertenza. Lo «smemorato di Detroit», come chiamo l'amministratore delegato Marchionne, fa riferimento a leggi di mercato, ma si tratta di leggi di mercato a metà, perché la FIAT in questi anni ha avuto da tutti i Governi

convochi immediatamente l'amministratore delegato della FIAT per risolvere questo problema. Oggi 18 dipendenti di una ditta dell'indotto di Termini Imerese sono stati licenziati, immediatamente, *d'emblée*, senza alcun tipo di preavviso, perché la FIAT ha deciso di far svolgere il servizio di ritiro